L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B ai Resoconti della seduta. Avverte

il provvedimento in esame, composto di un unico articolo ed approvato senza modificazioni alla Camera, dispone la conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 2011, n. 26, recante misure urgenti per garantire l'ordinato svolgimento delle assemblee societarie annuali, e consente di posticipare i termini della convocazione dell'assemblea annuale successiva alla chiusura dell'esercizio 2010 in favore di alcune tipologie di società quotate. Più in dettaglio, l'articolo 1, comma 1 del provvedimento, in deroga alle disposizioni vigenti, consente lo slittamento da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio 2010 dei termini per la convocazione dell'assemblea annuale anche qualora tale possibilità non sia prevista dallo statuto in favore di alcune tipologie di emittenti

investiti dell'obbligo di pubblicare alcune relazioni finanziarie a cadenza periodica (relazione finanziaria annuale, semestrale, resoconti intermedi di gestione). L'opportunità di consentire il predetto slittamento è motivata, secondo il Governo, dal fatto che le società sono tenute ad applicare le nuove norme Grazie, di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, apportando rilevanti modifiche alla normativa vigente in materia di interventi in assemblea e diritto di voto. Il comma 2 consente alle predette società, ove al 27 marzo 2011 (data di entrata in vigore del decreto-legge) abbiano già pubblicato l'avviso di convocazione dell'assemblea annuale, di convocare l'assemblea in prima o unica convocazione a nuova data. Il nuovo avviso deve rispettare i termini e le modalità di cui all'articolo 125-*bis* del TUF. L'assemblea deve pertanto essere convocata entro il trentesimo giorno precedente la data dell'assemblea stessa, con avviso pubblicato sul sito Internet della società e nel rispetto delle modalità dettate dalla CONSOB con regolamento. Nel caso di assemblea convocata per l'elezione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, il termine per la pubblicazione dell'avviso di convocazione deve essere anticipato al quarantesimo giorno I termini di convocazione di alcune particolari assemblee, convocate per riduzione del capitale sociale e per nomina o revoca dei liquidatori, sono spostati al ventesimo giorno precedente la data dell'assemblea. La nuova convocazione è possibile solo qualora non sia decorso, con riferimento all'assemblea originariamente convocata, il termine previsto nell'articolo 83-*sexies*, comma 1, del TUF, per l'invio delle comunicazioni che legittimano all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto nelle società italiane con azioni azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiana o di altri Paesi dell'Unione Europea con il consenso dell'emittente. Il comma 2 contempla altresì il caso in cui l'assemblea sia stata convocata anche per la nomina dei componenti degli organi societari. Viene anzitutto mantenuta anche per la nuova convocazione la validità delle liste già depositate presso l'emittente, con facoltà di presentarne di nuove nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 147-*ter*, comma 1-*bis*, del TUF, secondo il quale le liste sono depositate presso l'emittente entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet o con le altre modalità previste dalla CONSOB e dalle norme regolamentari emanate ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del TUF. La possibilità di rinvio a nuova data è estesa, infine, anche all'assemblea straordinaria convocata con il medesimo avviso.

Signora Presidente, l'ascolto della relazione del collega Mura mantiene l'esame di questo atto nei suoi Grazie,

come è noto a tutti, ed è inutile nasconderlo - una specifica situazione legata all'avvio di una catena di provvedimenti che ci fa dire che stiamo oggi assistendo alla prima puntata di una rappresentazione di cui abbiamo già visto la seconda puntata. Infatti, l'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011, che è poi la logica conseguenza

ha concesso dei tempi di recupero alla «nazionale imprenditoriale» italiana, che in questa partita è parsa francamente svogliata e distratta, e anche l'evoluzione odierna di questa partita ci conferma che una certa svogliatezza iniziale e distrazione vengono mantenute. Questo ci porta a riflettere su un problema storico del nostro sistema economico, un problema antico, perché il nostro è un sistema economico che vede un che vede un capitalismo senza capitali, che continua a non fornirci una risposta convincente ad una domanda strategica. Questo capitalismo senza capitali si è lasciato sfuggire l'occasione Parmalat, che pure era un'occasione estremamente interessante, perché era noto sul mercato che Parmalat aveva una grande liquidità interna che derivava dall'essere tornata vincitrice da una serie di contenziosi aperti con importanti banche rispetto alle vicende pregresse. Quindi, un'azienda risanata, un'azienda con grande liquidità, molto appetibile, e che fino al novembre-dicembre dello scorso anno era quotata 1,9 euro per azione, mentre oggi viene lanciata un'OPA da 2,6

noi abbiamo posto in essere, con tutte le criticità del caso, una serie di sbarramenti per impedire che questo avvenga, partendo dall'assunto che una Parmalat francese è sicuramente una perdita di valore per il nostro Paese; ma devo dire che anche il mantenimento in cattive mani di un'azienda italiana potrebbe essere una perdita altrettanto sgradevole. Come finirà questa operazione, quindi quale sarà il destino dell'applicazione di questo decreto, che è servito a guadagnare tempo e a consentire un tempo supplementare, oggi lo vediamo facilmente. Pare di capire che il tempo supplementare non è stato colto

difficilmente avrà concorrenti all'interno del nostro sistema, e la sospensiva ulteriore che è stata negata oggi dal TAR del Lazio ci fa sostanzialmente intravedere come si concluderà questa partita. lo sforzo fatto con questo provvedimento non è servito - noi l'avevamo detto anche nella discussione dell'articolo 7 del decreto n. del 2011 - a mettere in moto gli spiriti giusti dell'imprenditoria italiana, perché probabilmente una politica che è stata letta soltanto come una politica di difesa e non di attacco,

Quindi, non ha sortito l'elemento di acquisizione di fiducia del sistema produttivo e si è fermato al primo *step*, comprare tempo; il tempo è stato comprato, ma temo di dover dire - come ha scritto questa mattina su un noto quotidiano economico un brillante giornalista - «la frittata si può girare, ma pur sempre di frittata si tratta».

dal Presidente della Camera dei deputati il 4 maggio 2011, che è stato superato dai fatti. Quindi, a nostro giudizio, è un disegno di legge inutile. Quando si vuole difendere l'industria italiana acquisita

Intesa e Unicredit, che la fanno da padrone e decidono se, magari, devono salvare Alitalia

Voglio anche ricordare che noi ci troviamo di fronte a una Parmalat guidata da un signore di 82 anni, Enrico Bondi,

14 miliardi di euro del lattaio di Collecchio, 170.000 tra azionisti e obbligazionisti

non sappiamo quale sia il concetto di mercato per questo Governo e per questa maggioranza,

«Il numero uno di Parmalat, con il sostegno dell'intero consiglio d'amministrazione, alza l'ultima barricata contro l'assalto di Lactalis. "Il prezzo offerto dai francesi non è congruo", dicono da che è un prezzo non congruo? E quando Parmalat accumulava 1,4 miliardi di euro, senza accorgersi che questa azienda poteva essere contendibile, invece di rafforzarla e di impiegare queste risorse....

ha accumulato 1,4 miliardi di riserve, e quindi Lactalis compra Parmalat con tutte le conseguenze: e ciò dovrebbe preoccupare anche gli amici,

L'unica nota positiva per questo decreto è che Lactalis ha dovuto aumentare

Non voglio annoiare più di tanto, perché vedo poca attenzione in quest'Aula

noi dell'Italia dei Valori esprimiamo un giudizio molto severo su un decreto-legge che non serve a difendere l'industria nazionale

dovrebbe tutelare le ragioni del mercato e della concorrenza: quello è il giusto presidio per una nazione come l'Italia, e invece c'è una grande disattenzione rispetto a questo; forse ci accorgeremo che quello è il modo migliore per difendere i campioni nazionali.

Presidente, colleghe e colleghi, l'inutilità e l'irrilevanza del decreto‑legge che stiamo convertendo sono ormai acclarate, visto anche l'evolversi della situazione in queste settimane. un decreto confezionato con una motivazione burocratico‑legale generica, quella cioè di dare tempo alle società italiane di applicare le nuove regole del decreto legislativo n. 27 del gennaio 2010, con cui sono state recepite le direttive comunitarie, che risale quindi a ben 16 mesi fa. Se dovessimo fermarci a quella motivazione, dovremmo dire che questo decreto ci pone semmai di fronte ad un'ulteriore preoccupazione, legata all'incertezza giuridica che andrebbe a determinare. Il termine per la convocazione delle assemblee viene infatti affidato, anno dopo anno, all'iniziativa legislativa del Governo, magari attraverso il cosiddetto Perché introdurre questi elementi di discrezionalità in materia di diritto societario, una materia che ha invece bisogno di credibilità delle nostre regole, su cui regge la credibilità stessa dell'intero Paese? Tuttavia, il problema sotteso, e a tutti noto, che sta alla base delle scelte di questo decreto‑legge, riguardava il rinvio della convocazione dell'assemblea Parmalat per tentare di fermare l'acquisizione da parte di Lactalis:

perché il Governo, ancora una volta, ha voluto prendere una scorciatoia senza conoscere la meta e la direzione, o meglio, ha voluto improvvisare con un provvedimento privo di qualsiasi efficacia. Tutto questo non ha di certo celato, anzi evidenzi ancora di più la colpevole assenza di una politica economica ed industriale da parte del Governo. Sospeso tra dichiarazioni ondivaghe e contraddittorie (la scossa all'economia ferma da mesi al solo effetto annuncio, le frustate liberalizzatrici con la modifica dell'articolo 41 della Costituzione, l'intreccio tra spinte liberiste e, a giorni alterne, pulsioni nazionaliste), questo Governo non si è dato alcuna strategia per ridare fiato all'economia italiana. Anche perché, prima di decidere uno strumento, bisognerebbe decidere cosa fare, bisognerebbe essere in grado di prevedere e di programmare. Sta qui la discussione che dovremmo affrontare quando parliamo di italianità. Italianità come promozione di politiche, come visione lungimirante del ruolo e del posto del nostro Paese nelle dinamiche internazionali; italianità come forza del mercato interno che si confronta alla pari con il resto; italianità come una politica industriale che sappia coniugare vocazioni dei territori ed eccellenza dei settori; italianità insomma come capacità del sistema di offrire un ambiente favorevole per fare impresa, per rendere più competitivo il Paese, e quindi italianità come investimento in infrastrutturazione materiale ed immateriale, in ricerca, in formazione, in lavoro e nella sua qualità. Altro che italianità per decreto! Altro che italianità come difesa di un sistema debole e fragile! È per questi motivi che nel concetto di italianità rientra a pieno titolo la capacità di attrarre gli investimenti esteri, non certo di respingerli. Siamo il Paese che, in un confronto con gli altri Paesi europei, detiene la quota più bassa di imprese a controllo estero, il 4,1 per cento, meno della metà di quella francese e un terzo di quella del Regno Unito, come emerge da una recente ricerca in cui sono stati analizzati dati omogenei relativi alle imprese manifatturiere con almeno dieci addetti per sette Paesi europei. Certo che è corretto esigere reciprocità di trattamento e pretendere come Paese che a livello europeo le regole su questo tema siano rispettate e condivise; ma resta un dato di fatto incontrovertibile che il capitale estero rappresenti un'opportunità importante di crescita. I rappresentanti del gruppo Lactalis hanno precisato che il loro è un progetto industriale di crescita, volto allo sviluppo delle attuali aree di attività della Parmalat, sia in Italia che all'estero, con l'ambizione di diventare il principale operatore globale nel mercato del latte confezionato, nel rispetto delle realtà locali e in conformità alla propria vocazione industriale, conferma che valuterà l'opportunità di far confluire in Parmalat le proprie attività nel settore del latte, tra le quali quelle detenute in Francia e in Spagna, dando luogo così alla creazione di un campione di rilevanza mondiale, con sede, organizzazione e testa in Italia, in grado di confrontarsi con i maggiori operatori nazionali. È qui allora che entra a pieno titolo il ruolo del Governo: è fondamentale capire quali iniziative mette in campo per garantire che gli impegni dichiarati dal gruppo Lactalis diventino a tutti gli effetti impegni reali di sviluppo. Governo come intende valorizzare la filiera zootecnica italiana, quella lattiera-casearia in particolare, all'interno di questo campione mondiale del settore agroalimentare? Come intende valorizzare la qualità italiana di quel settore nel percorso di tutta la filiera e tutelare i produttori, anche in riferimento prezzo del latte, per non far sì che questo risulti indeboliti di fatto dal rischio di un sistema di monopolio? Colleghe e colleghi, ma quando e quanto in questi tre anni abbiamo avuto l'occasione di affrontare tali temi? Mai, nemmeno uno straccio di visione di politica per il Paese e per i suoi settori di eccellenza, non una misura a tutela delle imprese strategiche italiane. Parlando di filiera lattiero-casearia è persino imbarazzante constatare che lì, invece sì, una misura c'è stata, l'unica, quella vergognosa e reiterata della proroga del pagamento della multe sulle quote latte. È questo che intendete per italianità? Ancora una volta, come facciamo ormai da mesi, anziché discutere di tutto tranne che di politica industriale, il Gruppo del PD chiede che quest'Aula si dedichi finalmente a provvedimenti di natura organica, che si discuta seriamente sulla strategia industriale per il nostro Paese, che si discuta di politica economica, quella che determina le condizioni di sviluppo e di crescita del Paese.

finanze*. Rispondo ai colleghi affermando che si tratta di una normativa di portata generale, non occasionale, che introduce un elemento di flessibilità nell'attività di gestione delle società. Considerato che la convocazione delle assemblee dei soci delle società sarebbe una questione meramente tecnica, ci si riserva anno dopo anno, eventualmente tramite il decreto‑legge di proroga dei termini, il cosiddetto milleproroghe,

già approvato dal Senato e all'esame delle Camera dei deputati, ha autorizzato la Cassa depositi e prestiti ad assumere partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale

dare corso alle nuove leggi sulle reti, che sulla base di un libero contratto tra imprese consente la creazione di una entità consortile più grande, in grado di interloquire con banche, fisco e mercati da una posizione contrattualmente più forte. necessario ampliare l'ambito di operatività della Cassa depositi e prestiti come prima definito, al fine di accompagnare il processo di integrazione delle economie con un processo di crescita dimensionale, attraverso la disponibilità di risorse finanziarie e strumentali, *know-how* e nuove occasioni di lavoro. Pertanto, ritengo che questo provvedimento vada approvato, e condivido in pieno le osservazioni svolte dal relatore.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

trattarsi di un provvedimento di carattere generale che introduce elementi di flessibilità nell'autogoverno da parte del sistema delle società nell'approvazione di nuovi bilanci, l'emendamento è

si ritiene effettivamente di dover procedere ad elaborare una norma stabile. Il riferimento fatto dal Governo alla possibilità di intervenire nel decreto milleproroghe per prorogare il termine a 180 giorni è pertanto da considerarsi una misura assolutamente straordinaria, nel caso se ne verifichi la necessità. Sicuramente, c'è l'auspicio Grazie,

l'articolo 1, comma 1, del decreto‑legge, risultano assolutamente esenti da possibili azioni di responsabilità, essendosi - appunto - avvalsi

per consentire ad alcuni soggetti di approntare una difesa dall'acquisizione da parte dei francesi. Questo disegno di legge non servirà a nulla, poiché quasi sicuramente i francesi di Lactalis acquisiranno la Parmalat con i soldi di Parmalat, ossia 1,4 miliardi di euro, frutto di risarcimenti derivanti dal crack di 14 miliardi del «lattaio di Collecchio». Oggi, tutti si stracciano le vesti per difendere l'italianità, le imprese strategiche dall'assalto degli stranieri, mentre gli stessi erano distratti. Gli stessi che gridano oggi alla calata dei barbari e degli stranieri cercarono di favorire, meno di tre anni, fa il trasferimento di Autostrade: la gallina dalle uova d'oro che ottiene ogni anno consistenti incrementi tariffari a danno degli automobilisti, a prescindere dalla qualità dei servizi. Voglio ricordare che quel Ministro

è un disegno di legge inutile che offre, tra l'altro, molta discrezionalità nella gestione anche alla Cassa depositi e prestiti. Abbiamo visto quando c'è il potere discrezionale, senza controllo del Parlamento o pubblico, ciò che è accaduto in quei provvedimenti di protezione civile che hanno indotto alcune procure della Repubblica a rinviare a giudizio gli autori di quelle spese che erano state fatte, anche senza lo scrutinio della Corte dei conti. Per questa ragione, noi dell'Italia dei Valori voteremo contro un provvedimento inutile, che non risolve alcuno dei problemi.

Il Governo ha dimostrato in questa vicenda di non avere una visione complessiva di politica economica, men che meno industriale, e ha adottato provvedimenti soltanto episodici, volti a tamponare e a ricorrere a delle furbate. con questo provvedimento sia stato fatto un danno al Paese. Dobbiamo per un attimo ricordare - è già stata citata la vicenda Lactalis-Parmalat la Lactalis ha fatto un'operazione di acquisizione del 29 per cento delle azioni di Parmalat, investendo circa un miliardo di euro che le avrebbero consentito di avere il controllo del consiglio di amministrazione.

e, quindi, di non dare il segnale che le regole si possano cambiare secondo le convenienze o gli umori: occorrono bensì regole certe, che possano

L'Italia non ha bisogno di provvedimenti tampone o soltanto di tipo conservativo, ma di provvedimenti di sviluppo della sua economia, quindi di una politica industriale di ampio respiro e di decisioni accorte, accorte, anche estese, di politica fiscale. Le aziende devono essere stimolate e incentivate. Gli imprenditori che decidono di investire e di rischiare devono essere garantiti ed agevolati. Per queste considerazioni,

Signora Presidente, gentili membri del Governo, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 26 nasce dalla necessità di dare una pronta risposta alle aziende del nostro Paese, nel tentativo di fermare la scalata al capitale e alla gestione dei nostri maggiori colossi da parte di aziende straniere. Con il decreto-legge in esame viene data la possibilità all'organo amministrativo delle società di rinviare lo svolgimento dell'assemblea ad una data che può arrivare fino al 30 giugno, dando in tal modo la possibilità ad altri gruppi industriali, magari nazionali, di formare cordate alternative garantendo importanti settori del nostro sistema economico. Il decreto nasce sicuramente dalla necessità di intervenire rispetto alla scalata partita nelle scorse settimane con l'acquisizione, diretta o indiretta,

con questo decreto-legge viene data la possibilità ad altri gruppi industriali di formare cordate alternative. La proposta più rilevante, anche oggi in Aula, è stata sicuramente quella di rendere permanente le disposizioni di di questo decreto-legge, posticipando in maniera definitiva il termine per la convocazione dell'assemblea a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. A questo credo di aver già risposto prima in termini di parere sugli emendamenti. Sicuramente, una scalata sul tipo di quella avviata nei confronti della Parmalat deve essere contrastata con strumenti non solo legati a norme giuridiche nazionali ma per lo più a norme comunitarie, e quindi deve essere contrastata nelle sedi appropriate nelle quali gli interessi degli Stati dovrebbero essere reciproci e non di pura convenienza di uno Stato rispetto ad un altro. La Lega Nord ha sempre ribadito l'importanza del sostegno non soltanto ai grandi gruppi industriali ma anche ai piccoli e ai medi che operano in settori strategici, e il settore alimentare è sicuramente uno di questi. Si tratta infatti di un settore il cui indotto coinvolge numerosi piccoli allevatori e una miriade di imprese agricole di tutte le dimensioni. Mantenere quindi la *governance* significa avere le basi necessarie per un polo lattiero-caseario di livello internazionale. Voglio sottolineare quanto sia necessario introdurre principi che pongano le nostre società al riparo dall'acquisizione da parte di società estere, quando in altri Paesi esistono norme a tutela delle rispettive società ed economie. Ritengo che nel 2007, in sede di discussione della legge 20 giugno 2007, n. 77, che recepiva la direttiva europea in termini di OPA, al Governo Prodi siano forse mancati il coraggio, la capacità politica o la forza di incidere su una direttiva europea che avrebbe dovuto tenere conto di quegli aspetti fondamentali per il futuro del nostro sistema economico. La Lega Nord è assolutamente a favore del libero mercato, ma con regole chiare per tutti. all'epoca, aveva combattuto una battaglia perché vi fossero norme in grado di tutelare efficacemente gli interessi delle nostre società, come avveniva in molti altri Stati che avevano infatti stabilito garanzie a favore delle loro imprese oggetto di offerte pubbliche. Oggi non si può ancora sapere come evolverà definitivamente la situazione Parmalat: riteniamo però che il Governo, con questo provvedimento, abbia agito con assoluto senso di responsabilità e si sia mosso per tutelare, con queste e con altre norme, le nostre aziende anche di fronte all'Unione europea, che spesso dimostra fragilità e poca omogeneità nella definizione delle regole del gioco. Ho già detto del rammarico di aver perso del tempo utile per gettare anche le basi di un'effettiva tutela della nostra economia; non si è voluto dire nulla, arrivando però oggi a questo provvedimento che posticipa i termini di 60 giorni e dà la possibilità - ribadisco ancora una volta - a eventuali soggetti italiani di formare in grado di tutelare le nostre aziende, non soltanto quindi Parmalat, ma altre eventuali nostre imprese in settori importanti della nostra economia. pertanto che questo provvedimento sia sufficiente per provare a non disperdere un nostro grande patrimonio, e con questo annuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord.

come abbiamo ascoltato, il Governo ha detto che questa è una norma di portata generale; l'ha invocata con la motivazione della necessità per le società di assorbire meglio le novità previste in sede di prima applicazione del decreto legislativo adottato nel gennaio del 2010. In questo modo, ha fatto torto all'immagine e alla capacità delle società interessate, come se quindici mesi non fossero un tempo sufficiente per uniformarsi a quelle novità normative. Del resto, basterebbe scorrere molte cronache (anche di colore, per la vivacità dei dibattiti, la partecipazione e la novità dell'esercizio del voto in forma telematica) che hanno accompagnato le tante assemblee societarie che si sono svolte nel corso di queste ultime ultime settimane, per dimostrare l'infondatezza di questo assunto. Se poi si intendeva introdurre una misura ordinaria di maggiore agio per favorire lo svolgimento delle assemblee e la partecipazione degli azionisti, non si sarebbe dovuto dovuto rigettare l'emendamento che avevamo presentato per una modifica del codice civile. Tra l'altro, voglio ricordare che, avendo l'Assemblea oggi detto di no a questa norma, a vedere introdotte nei prossimi milleproroghe, così ha detto il Ministro dell'economia alla Camera, norme annuali che attivino o neghino - a suo invece che regole per tutti, discrezionalità e arbitrarietà, come se spostare le assemblee già convocate e l'incertezza in tema di scadenze da rispettare fosse un modello da auspicare piuttosto che l'eccezione da cercare di evitare. In realtà, questo decreto, come è stato detto con onestà intellettuale dal relatore, è stato approvato proprio allo scopo di intervenire sulla vicenda Parmalat, perché mi risulta che solo altre tre società se ne siano avvalse e per motivi del tutto diversi.

però, nella sua ipocrisia e anche nella sua patente inefficacia rispetto alle intenzioni che lo sorreggevano, esso è un paradigma dell'inadeguatezza e dell'incapacità dell'azione di questo Governo. infatti certo che ci sarebbe bisogno di curare e potenziare la filiera produttiva del latte, quella dell'agro-alimentare e più complessivamente il comparto agro-industriale, ma per questo ci vorrebbe una politica industriale, non provvedimenti estemporanei e controproducenti. che Parmalat potesse essere un oggetto interessante e appetibile sul mercato non era cosa sconosciuta: già da gennaio - cito fonti CONSOB hanno iniziato a circolare indiscrezioni circa possibili iniziative da parte di grandi investitori internazionali presenti nel capitale di Parmalat, in vista della prossima scadenza del consiglio di amministrazione. Non si poteva fare qualcosa prima, invece che aspettare fine marzo? Ma in quel mese, gennaio, il Governo si trastullava con il processo breve e con qualche favore ai soliti noti con il rinvio delle multe sulle quote latte. In questo c'è drasticamente la raffigurazione della siderale distanza tra i l'azione del Governo e i problemi del Paese, perché o ci si occupa di tutt'altro o ci si accontenta di guardarsi la punta delle scarpe.

Scontiamo l'assenza di una politica industriale in grado di coniugare vocazione dei territori ed eccellenze dei diversi settori produttivi dunque, quando le imprese dicono di sentirsi lasciate sole e i lavoratori lamentano la mancanza di una politica per la crescita e l'occupazione hanno ragione.

Ci sono stati diversi episodi che hanno messo a nudo la nostra debolezza, che hanno evidenziato le responsabilità e l'assenza di capacità di azioni in positivo del Governo? Basta costruirsi un nemico, invocare l'italianità e provare in questo modo a costruire un manifesto di intenzioni abbastanza suggestivo in grado di costruire un consenso a breve, salvo poi andare alla verifica dei risultati effettivamente conseguiti.

e, soprattutto, chi volesse investire dall'estero probabilmente non sarebbe motivato. Insisto su questo tema. Noi siamo per la difesa dei valori, del patrimonio e delle capacità produttive del Paese, ma attenti a non demonizzare gli investimenti che vengono dall'estero. Ne abbiamo bisogno, siamo sotto la media europea, abbiamo necessità di elementi che apportino capacità, valore, possibilità di occupazione e di innovazione. Per questo, quindi, è necessaria una politica industriale. Al collega Mura dico:

proposito, va bene mettere a disposizione risorse per sostenere la capacità di rafforzamento del sistema produttivo anche con interventi pubblici, ma non possono essere affidati alla discrezionalità del Ministro dell'economia che può decidere a suo piacimento su quale impresa far confluire risorse pubbliche. Ci vogliono investimenti che vadano ad incidere sui fattori strutturali, sugli elementi di competitività del sistema, sulla ricerca, sull'innovazione, sulle infrastrutture, sulla politica energetica. Se non si fanno queste cose si crea una situazione di assoluta inefficacia degli interventi, anche solo dal punto di vista della salvaguardia degli interessi che dovremmo presidiare, e cioè la filiera, l'occupazione, i piccoli risparmiatori, l'interesse dei consumatori.

che il Governo verificasse effettivamente l'affidabilità di quel piano industriale. Insomma, questi elementi dimostrano che c'è stata approssimazione, che questo provvedimento in realtà non ha prodotto niente all'effetto che voleva conseguire, se non una brutta figura, in termini complessivi e generali, per il Governo e per il Paese. Questo chiama in causa il fatto che bisogna discutere diversamente di una politica industriale. Sono anni anche nelle ultime settimane) che vi sollecitiamo a discutere di politiche industriali per il rilancio della crescita e per lo sviluppo e l'aumento dell'occupazione. Su questo ribadiamo la disponibilità ad un confronto e, visto come stanno andando alcune tendene che si muovono nel Paese, forse vi converrebbe tenere più conto delle nostre sollecitazioni e affrontare finalmente una discussione seria e di merito, non solo per il rigore dei conti ma anche per il sostegno della crescita.

Signora Presidente, non urlerò, non ce ne sarà bisogno, perché sarò senz'altro breve e sintetica nel dichiarare il voto favorevole del Popolo della Libertà alla conversione in legge del decreto-legge in esame, che consente di posticipare da 120 a 180 giorni il termine per l'approvazione dei bilanci 2010 in favore delle società quotate. Una disposizione di cui nella prossima stagione assembleare, che stiamo già vivendo

è francamente non consono a chi sta svolgendo una dichiarazione di voto, come lei fa notare tutte le volte che interviene. Una disposizione di cui nella prossima stagione assembleare, che stiamo già vivendo in queste settimane, potranno avvalersi le società toccate dal recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva n. 36 del 2007. La norma infatti fa riferimento all'articolo 2364 del codice civile - che hanno più volte citato i colleghi che mi hanno preceduto - innovato lo scorso anno, che già prevede la possibilità di convocare, non oltre 180 giorni, l'assemblea per quelle società tenute alla redazione di bilanci consolidati ovvero per particolari e motivate esigenze relative all'oggetto e alla struttura di quelle società. Da questo punto di vista, le disposizioni del decreto-legge intendono rendere strutturale la norma possibilmente in un insieme normativo di livello europeo, affinché la regola sia rispettata in tutti gli Stati dell'Unione europea, con il fine di evitare quanto già accaduto precedentemente a scapito di scalate messe in atto, per esempio, dalle nostre aziende: questo era quanto ha affermato il Ministro dell'economia ed il Governo in sede di discussione alla Camera. discussione alla Camera. A proposito dell'ipotesi che la reiterazione di questa norma e la sua conferma anche per il prossimo bilancio possa avvenire nel milleproroghe, noi la pensiamo la pensiamo diversamente dal senatore Barbolini: pensiamo che forse, prima ancora del milleproroghe, alla luce degli esiti che verranno generati dall'applicazione di questa norma, in questa fase e in questa tornata di assemblee societarie, potremmo svolgere una riflessione più approfondita e precisa, valutare quante società hanno davvero utilizzato e colto l'opportunità di utilizzare l'ampliamento dei termini e decidere se valga la pena oppure no confermare questa norma. Questo è però un aspetto tecnico, che apre il campo a riflessioni non tecniche. Infatti, abbiamo assistito a polemiche, scambi di opinioni giornalistiche, fondate sostanzialmente sull'idea che con il provvedimento il Governo era intenzionato a difendere l'italianità di aziende sottoposte ad attacchi proprietari da colossi dell'Oltralpe; è il caso specifico di Parmalat e Lactalis, che stiamo evocando

dell'agroalimentare, ad esempio - che, seppure importantissime, mi sembra però non siano ancora beni pubblici e, quindi, oggetto di un particolare interesse di natura pubblica, come il comparto dell'energia. L'iniziativa assunta dal Governo non è in funzione antiscalata: intende dare agli amministratori, in questo caso della Parmalat, ma più in generale a tutti coloro che si trovano o si troveranno in questa situazione, il il tempo necessario per verificare, cosa che infatti Parmalat sta facendo, in attesa dello svolgimento dell'assemblea annuale, l'esistenza di eventuali ipotesi alternative di acquisizione, che siano più o meno vantaggiose - noi ci auguriamo sempre di più - per gli azionisti. La storia di Parmalat - non la voglio ricordare in questo momento perché ruberei troppo tempo all'importante dibattito dell'Aula - è costellata di prese di posizione, anche di tipo giudiziario, che hanno sollevato un'attenzione particolare e quindi la necessità che il Governo e la maggioranza che lo sostiene siano su questo caso particolarmente attenti; non è infatti nostra, ma della procura della Repubblica l'iniziativa di approfondire e indagare su alcuni passaggi evidentemente poco chiari. Quindi, si tratta - come più correttamente ha sostenuto il senatore Cantoni - di dare un segnale di una corretta politica di *corporate governance* - come dicono i grandi esperti - nei confronti quel momento avrebbe voluto aggirare l'obbligo di OPA da fondi speculativi esteri per consegnare il controllo di una società quotata in borsa ad una non sottoposta ai vincoli, alle tutele e agli azionisti - quelli, che sono molto cari al senatore Lannutti - nel percorso di acquisizione di una società importante come Parmalat, che sappiamo tutti detenere uno straordinario tesoretto nelle sue casse, frutto dell'oculata amministrazione di questi anni. Quello che ci Quello che ci accingiamo ad approvare non è tanto uno strumento protezionista: è un mezzo per dotare l'Italia di norme simili a quelle presenti in altri Paesi, che consentono di determinare comportamenti anticoncorrenziali, da poteri poteri dominanti di qualsivoglia natura. È un atto che in qualche modo possiamo considerare dovuto, volto paradossalmente a rafforzare la logica delle regole di mercato - e non di protezione - vigenti in ambito nazionale e comunitario, soprattutto basate su quel principio di reciprocità che regola tutti i buoni mercati.

del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, recante misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia,

Onorevoli colleghi, stiamo passando al punto successivo all'ordine del giorno, che prevede la relazione del relatore e una serie di interventi, però non in questo frastuono. Vorrei pregarvi di non obbligarmi a sospendere la seduta.

il decreto-legge all'esame dell'Assemblea dispone l'erogazione di 345 milioni di euro, per il triennio 2011-2013, in favore del personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale e della Polizia penitenziaria. Nello specifico, il comma 1 dell'articolo 1 prevede che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, la dotazione del fondo del medesimo decreto-legge sia incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro. L'articolo 8 del decreto-legge n. 78 del 2010 ha istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2011 e 2012, destinato al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco interessato dal dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali, disposto dall'articolo 9, comma 21, dello stesso decreto-legge n. 78 del 2010. A seguito dell'intervento disposto dal decreto in esame,

non solo disporrà di 115 milioni di euro in più per ciascun anno del biennio 2011-2012, ma diventa triennale, con una dotazione di 115 milioni anche per il 2013. Il comma 2 prevede la possibilità di una successiva ulteriore integrazione del citato fondo per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Il comma 3 stabilisce inoltre che il fondo per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico sia destinato alla corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

della spesa di cui ai commi 1 e 21 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 78; dall'altro lato, fa riferimento al personale interessato al riconoscimento di una serie di benefici economici (assegno funzionale; trattamento economico superiore correlato all'anzianità di servizio senza demerito, compresa quella nella qualifica o nel grado; incrementi stipendiali parametrali non connessi a promozioni; emolumenti corrispondenti previsti per i Vigili del fuoco). Il provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni riunite affari costituzionali e difesa in due sedute che si sono svolte in questi giorni. Non sono stati approvati emendamenti, ma è stato accolto dal Governo un ordine del giorno, presentato dal senatore Saltamartini, che ringrazio per averlo presentato, al quale hanno aggiunto la loro firma i senatori di maggioranza e di opposizione delle due Commissioni. Il tema, d'altra parte, non poteva non essere condiviso da tutte le forze politiche che responsabilmente hanno a cuore le esigenze del comparto sicurezza e difesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la funzione fondamentale che esso svolge a tutela della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico. Dal momento che tale comparto era stato interessato dal blocco retributivo previsto dal decreto-legge n. 78 del 2010, con l'ordine del giorno accolto si impegna il Governo a intraprendere ogni idonea iniziativa volta a prevedere il mantenimento in bilancio delle eventuali somme residue del fondo perequativo per gli anni 2011, 2012 e 2013, anche a incremento delle dotazioni stabilite per i medesimi anni, nonché a consentire l'utilizzo delle stesse somme non impegnate o non impiegate nell'anno precedente anche attraverso modalità attuative da definire con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

battono il territorio del nostro Paese per garantire la sicurezza dei cittadini e combattere la criminalità organizzata, il riconoscimento del loro lavoro, mettendo a disposizione queste risorse, che rappresentano certamente solo una parte di quello che avremmo dovuto fare, ma una parte importante, perché è l'inizio di un processo che il Governo saprà portare avanti.

ha già svolto nelle sue parti fondamentali la relazione sul disegno di legge n. 2716, al quale noi diamo grandissima importanza per sottolineare l'attenzione del Governo e della maggioranza, ma in linea generale - noi riteniamo - di tutta l'Assemblea, in favore del personale del comparto sicurezza, la cui specificità è da anni oggetto di riconoscimento legislativo.

che mai come in questi ultimi anni il Governo Berlusconi ha portato avanti, secondo un concetto di attento e severo controllo della malavita. del 2011, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, come è già stato detto, prevede uno stanziamento di 345 milioni.

La disposizione riformulata conferma la possibilità di incrementare ulteriormente il fondo, sia a seguito delle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace, sia con una quota parte di quanto destinato al fondo unico giustizia, stabilendo, altresì, che l'attribuzione delle predette risorse, globalmente intese, deve assicurare trattamenti omogenei al personale delle Forze armate e a quello delle Forze di polizia. Il testo originario della norma prevedeva, invece, che gli assegni per il personale militare fossero finanziati esclusivamente con i proventi derivanti dalle minori spese per le missioni internazionali, indirizzando conseguentemente la quota derivante dal fondo unico giustizia agli assegni per il personale delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. Nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite

presidente Vizzini - è stato accolto dal Governo ed impegna l'Esecutivo a intraprendere iniziative volte al mantenimento in bilancio delle somme residue del fondo perequativo per gli anni 2011, 2011, 2012 e 2013. È un disegno di legge che fa onore alla nostra Assemblea, e del quale siamo estremamente orgogliosi. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Del Vecchio. Ne ha facoltà. il disegno di legge che oggi esaminiamo è relativo ad una tematica di notevole importanza, in quanto attiene alla equilibrata e funzionale operatività delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo dei vigili del fuoco. Tre comparti a cui il nostro Paese affida compiti delicatissimi e primari, quali il controllo del territorio nazionale, la sicurezza interna ed esterna, la salvaguardia delle istituzioni democratiche, gli interventi in occasione delle pubbliche calamità, la lotta alla criminalità. Tre comparti, quindi, che chi è chiamato al governo del Paese non può non considerare strategici per la vita della Nazione, per la serenità dei cittadini e per il rispetto degli accordi e delle alleanze. Proprio per questi motivi, per l'importanza delle funzioni della sicurezza e della difesa, erano state accolte con grande stupore da parte dei cittadini le le misure riduttive che questo Governo aveva adottato nel 2010 nei confronti delle retribuzioni del personale appartenente ai comparti in argomento. Stupore da parte dei cittadini, dicevo, ma anche disagio morale nei destinatari di quel provvedimento - il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia dei Vigili del fuoco - che non riuscivano a comprendere, e tuttora non comprendono, lo stridente contrasto tra il riconoscimento e l'esaltazione della loro funzione e della insostituibile opera che svolgono, espressi continuamente anche da esponenti importanti del Governo e della maggioranza, e la penalizzazione che questo Governo ha posto in atto nel 2010 alle loro già scarse retribuzioni. Per queste ragioni, per le giustificate reazioni negative a quel provvedimento, va accolto con favore il fatto che l'Esecutivo ha finalmente compreso la necessità di rivedere le decisioni assunte nel 2010. D'altro canto, il Parlamento, in più circostanze nell'ultimo anno e con numerosi ordini del giorno, ha sollecitato il Governo ad operare per sanare gli inconvenienti che si sono determinati. Purtroppo, però, il giudizio nei riguardi dell'iniziativa dell'Esecutivo non può essere positivo nella misura in cui sarebbe stato auspicabile. Il provvedimento che viene proposto, infatti, non elimina gli effetti degli ingiustificati tagli alle retribuzioni del personale in argomento; addirittura, prevede aspetti ancora penalizzanti per gli operatori dei tre comparti. Innanzitutto, le risorse finanziarie destinate alle misure perequative appaiono insufficienti. Il personale in argomento ammonta complessivamente a più di 400.000 unità e, pur nella diversità delle perequazioni da attivare e da calcolare caso per caso, gli assegni da elargire avranno un importo medio di 25 euro: cifra, direi, assolutamente irrisoria. Sarà quindi necessario integrare sensibilmente il fondo per le perequazioni nell'anno in corso ed in quelli che seguiranno, con particolare riferimento al 2013, allorché non sarà disponibile l'aliquota di 80 milioni di euro, prevista solo per il 2011 e il 2012. Un secondo aspetto del provvedimento non in armonia con le aspettative del personale è quello relativo alla natura delle misure perequative. Sorprendentemente, il Governo ha deciso di attribuire alle misure in argomento le caratteristiche di *una tantum* e non le ha considerate, come invece era lecito attendersi, assegni individuali aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento che dovrebbero sostituire. Ciò determinerà evidentemente penalizzazioni nel settore previdenziale a carico del personale in questione. È evidente, quindi, come gli aspetti di cui ho parlato - la limitatezza delle misure perequative predisposte dal Governo, la natura di queste stesse misure - siano in contrasto con il riconoscimento dovuto della peculiarità dell'impiego e del ruolo delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: quella specificità che il Parlamento ha finalmente riconosciuto al personale dei tre comparti proprio in questa legislatura. In sostanza, mentre con dichiarazioni in circostanze particolarmente difficili vengono esaltati il senso di sacrificio, lo spirito di servizio, la pronta disponibilità del personale in argomento, mentre frequentemente si riconoscono i suoi obblighi e le limitazioni previste da leggi e regolamenti o si esprimono nei suoi riguardi apprezzamento e riconoscenza per quanto fa continuamente, poi, in un momento così importante come quello del disegno di legge all'esame, il Governo purtroppo non riesce ad assicurare pienamente ciò che non può essere considerato un privilegio, bensì il giusto riconoscimento dell'impegno di quelle categorie di servitori dello Stato. Sembra al riguardo che il Governo abbia perseguito in questa circostanza l'intendimento di promuovere un provvedimento parziale e limitato e non abbia operato per sviluppare una politica di forte supporto ai comparti della sicurezza e della difesa. Sottolineo ancora un altro aspetto del provvedimento che necessita - a mio modo di vedere - di una sostanziale modifica. Le risorse per la corresponsione degli assegni *una tantum* al personale di cui stiamo trattando verranno tratte da quelle accantonate per il riordino delle carriere nei tre comparti. È un colpo forse definitivo alle speranze di quel personale di vedere realizzata una riforma di sistema - il riordino delle carriere - assolutamente urgente e dallo stesso personale, da tutto il personale, continuamente sollecitata. Concludendo, credo di poter affermare che il provvedimento all'esame è l'occasione per una reale e concreta dimostrazione di attenzione nei confronti di una categoria stimata e apprezzata da tutti. Lo scopo è stato raggiunto solo in maniera parziale e, certamente, non come quel personale si attendeva. È una occasione che il Governo non ha colto appieno, ma che potrebbe dare comunque un esito positivo qualora fossero accolte le proposte che il Partito Democratico formulerà in sede di esame degli emendamenti, e che riguarderanno proprio gli aspetti negativi che ho evidenziato.

marzo 2011, n. 27. Questo provvedimento reca misure urgenti per la corresponsione di assegni *una tantum* al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Peccato si tratti solo ed esclusivamente di qualcosa che era stato tolto ingiustamente ai militari, solo qualche mese addietro, e che, per compiacere il ministro Tremonti, non si restituisce in modo definitivo, come si sarebbe dovuto fare, ma *una tantum*. Infatti, colleghi, al comma 1 dell'articolo 1 si prevede che, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 ed in particolare dai commi 1 e 21 del predetto articolo (ovvero il blocco degli scatti), la dotazione del fondo di cui all'articolo 8, comma 11-*bis*, del medesimo decreto-legge sia incrementata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, di 115 milioni di euro. Vorrei ricordare al riguardo, infatti, che la normativa oggi vigente - quella che la maggioranza ha approvato nel 2010, convertendo l'ennesimo decreto di finanza creativa tremontiana, il decreto n. 78 - ha bloccato, per il triennio 2011-2013, il trattamento economico individuale complessivo dei dipendenti pubblici, anche di qualifica dirigenziale, prevedendo che esso non possa in ogni caso superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010. Questo significa, colleghi, per dirla in parole povere, che i capitani possono pur diventare colonnelli, ma continueranno ad essere retribuiti da capitani. Non solo. Come saprete, sempre lo stesso decreto, all'articolo precedente a quello che introduceva il blocco degli scatti - ovvero all'articolo 8 ha disposto l'istituzione di un fondo destinato - leggo testualmente - «al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» interessato dal blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli automatismi stipendiali, disposto dall'articolo 9. Questo fondo, per il triennio 2011-2013, aveva come dotazione 80 milioni di euro. Ora, con il decreto in esame gli si aggiungono 115 milioni di euro annui. Occorre ricordare che si tratta non di una aggiunta dovuta alla magnanimità del Governo o di questa maggioranza, ma semplicemente di una necessaria aggiunta perché i fondi già individuati - gli 80 milioni di cui sopra - sono già esauriti. Ciò detto, e continuando con il decreto in questione, al comma 2 dell'articolo 1 è stabilito che la dotazione del fondo possa essere incrementata - anche qui leggo testualmente «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze(...) con quota parte delle risorse corrispondenti alle minori spese effettuate, rispetto al precedente anno, in conseguenza delle missioni internazionali di pace, e delle risorse di cui al comma 7, lettera *a)*, dell'articolo 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 (...), relativo al Fondo unico giustizia». Ci troviamo, quindi, davanti a un'autorizzazione che il Parlamento dà al Ministro dell'economia per spostare eventuali fondi risparmiati da altre amministrazioni dello Stato - quali il Ministero della giustizia o il Ministero della difesa - per incrementare il famoso fondo *una tantum*. Cioè, praticamente, colleghi, si dice: vorremmo darvi di più perché sappiamo che questi soldi son pochi e non bastano neppure per un semestre, ma autorizziamo ad aumentare detto contributo con i soldi che dovessero avanzare dalle missioni internazionali o dal Fondo unico giustizia. A questo punto, colleghi, c'è davvero qualcosa che non mi torna! Come ben sappiamo, i soldi non bastano mai per nessuna Amministrazione dello Stato, figuriamoci per le onerosissime missioni internazionali che ci troviamo a rifinanziare puntualmente ogni sei mesi. Figuriamoci anche l'effetto di questo provvedimento sulla giustizia, con i tanti e gravissimi problemi da cui essa è afflitta. Problemi che emergono soprattutto a causa della scarsità dei fondi e non, come invece questo Governo vuole farci intendere, esclusivamente dalla cattiva amministrazione degli stessi e dalle *défaillances* strutturali del sistema. Non è riformando il sistema giustizia che possiamo risolvere questi problemi. Diamo loro i fondi che invece intendiamo persino togliere e vedremo come la durata dei processi diventerà ragionevole senza ledere i diritti di alcuno. Tornando al decreto-legge in esame, il Governo, che puntualmente dice di non avere i soldi per finanziare a dovere le missioni internazionali e il Fondo unico giustizia, ci dice oggi che in futuro, se queste spese dovessero magicamente ridursi, Tremonti potrà trasformarle in aumenti di stipendio *una tantum* - mi verrebbe da dire «*una paucum*» - per gli ufficiali. È di questo che stiamo parlando? Ma vi sembra forse un modo di costruire la legislazione dello Stato? A questo punto, segnalo anche un forte timore, di fronte ad ulteriori atti normativi - oltre a quelli che normalmente discutiamo, si intende - con i quali finanziare i fondi delle missioni internazionali e il Fondo unico giustizia. Nutro il sospetto che questo possa essere stato voluto di proposito al fine di far avanzare detti finanziamenti e che questi siano quindi spostabili dal ministro Tremonti su altri capitoli, facendo intanto credere oggi ai militari che gli stessi soldi potrebbero essere destinati a loro. La memoria corre al ventennio fascista, quando gli armamenti venivano trasferiti da un posto all'altro in occasione delle visite del duce per far credere che la dotazione fosse composta da un elevatissimo numero di unità, per far moltiplicare fittiziamente le poche risorse a disposizione. Non è altro che un tranello finanziario! Un gioco delle tre carte! Tutto ciò, colleghi, risparmiandovi i dettagli sulle norme oggi in vigore e sulle modalità di assegnazione dei soldi di cui al Fondo unico per la giustizia. Sottolineo invece che, supponendo che le economie di spesa sulle missioni internazionali e sul Fondo unico per la giustizia si realizzino, l'eventuale incremento del fondo le cui risorse finanziano gli interventi previsti dal decreto-legge in esame andrà disposto con decreto ministeriale. L'intervento non risulterebbe quindi sottoposto alle consuete procedure di verifica parlamentare dei profili di carattere finanziario. Inoltre - leggo testualmente una parte della nota del Servizio studi della Camera dei deputati «non sono esplicitate le modalità di accertamento e riassegnazione dei predetti risparmi: non risulta quindi possibile verificare se le stesse siano idonee, per un verso, ad evitare che le somme in questione vadano in economia e, per altro verso, a garantire un utilizzo entro termini coerenti con le precedenti previsioni di impiego, al fine di evitare disallineamenti sul piano temporale, con conseguenti effetti di cassa. Sul punto appare necessario acquisire una valutazione del Governo». In proposito, occorre considerare che i provvedimenti di finanziamento delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia prevedono attualmente stanziamenti di durata semestrale. Passando ad analizzare il comma 3, dell'articolo 1, emerge con chiarezza la confusione che avvolge questo provvedimento e l'intenzione subdola del Governo. Si parla, infatti, di corresponsione di assegni perequativi individuali, aventi la stessa natura dell'emolumento corrispondente, che nel titolo sono stati definiti *una tantum* e che altro non sono che sacrosanti aumenti di stipendio dovuti all'avanzamento del grado, cioè qualcosa che andrà elargita mensilmente, quanto meno per i tre anni che ci si è preoccupati di finanziare con questo decreto, mantenendo, però, in vigore il blocco degli scatti. È veramente pura demagogia. Ma non è finita qui, colleghi. Al comma 4 è contenuta la copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma 3 in questione. Lì si dispone che alla copertura finanziaria si provveda «mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2011, 2012 e 2013, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 Tale ultimo periodo autorizzava, tra l'altro, la spesa di 122 milioni dì euro, a decorrere dall'anno 2006, da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Quindi, per completare il capolavoro dell'ingiusto ed iniquo taglio degli scatti stipendiali, prima glielo si ridà *una tantum*, ma mantenendo il taglio stesso, e poi, per coprire la marachella, cosa si fa? Si tagliano i fondi da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Si potrebbe dire che, all'interno di una guerra tra poveri, si toglie ai più poveri per dare ai meno poveri. Vedete, colleghi, e concludo, l'Italia dei Valori non può essere contraria ad una norma con la quale si restituiscono soldi ai militari, soldi questi ultimi, colleghi, vogliate perdonare la terminologia, fregati loro con precedenti atti che la maggioranza ha adottato. Ma, al contempo, non ci si può chiedere di avallare una simile legislazione e non ci si può chiedere di accettare che i soldi che si restituiscono agli uni vengano tolti a settori che ne avrebbero altrettanto bisogno.

alle risorse operato con il decreto Tremonti, al fine di scongiurare la palese incostituzionalità derivante dal blocco dei benefici economici legati all'avanzamento in qualifica, utilizza le risorse allocate ed accantonate per l'anno in corso e relative al riordino delle carriere al fine di attribuire un emolumento perequativo in luogo del blocco dei benefici economici legati all'avanzamento in qualifica. Tali risorse, aggiunte agli 80 milioni già stanziati per sopperire al medesimo meccanismo introdotto dallo stesso decreto Tremonti, sono state sufficienti a coprire tutte le esigenze dell'intero comparto sicurezza e difesa, Vigili del fuoco compresi, anche contabilizzando i riflessi economici necessari per garantire la copertura ai fini previdenziali della buonuscita, per il solo anno 2011. È opportuno sottolineare che la medesima soluzione, anche con effetti ai fini previdenziali di buonuscita, è già stata operata altre due volte sul comparto Sicurezza e Difesa: la prima volta nel 1995, a seguito del riordino delle carriere operato in quell'anno; la seconda volta nel 2003, quando vi fu una norma che trasformò i livelli stipendiali in parametri stipendiali con l'applicazione della legge n. 153 del 2003. Per cui, è assolutamente infondata l'obiezione del Ministero dell'economia sull'impossibilità a praticare una soluzione di questo tipo. Ma l'aspetto veramente incredibile risiede nel fatto che il Governo, proprio per evitare opposizione e strumentalizzazione da parte dello stesso Ministero, aveva garantito gli emendamenti, prima approvati in Aula a Montecitorio, poi cassati per effetto del parere contrario della Commissione bilancio.

di ridurre al minimo i danni e le mortificazioni che gli uomini e le donne che vi operano subiscono ormai da anni. In ultimo, si sottolinea che per il 2012 mancano circa 85 milioni per effettuare la stessa operazione. Lo stesso avviene per il 2013, laddove la somma ammonta a 185 milioni, quali, come originariamente previsto, dovevano essere reperiti dai fondi per la riduzione delle missioni all'estero per quanto riguarda le Forze armate, mentre per le Forze di polizia dal Fondo unico per la giustizia. Il non voler riconoscere questa opportunità, cioè consentire che le proprie risorse possano sanare anche l'aspetto previdenziale e gli effetti sulla buonuscita, rappresenta una mortificazione per chi, come le donne e gli uomini del comparto Sicurezza e Difesa, opera quotidianamente con risultati di grande eccezionalità. Sarebbe stato invece preferibile estrapolare una strategia lungimirante, per sostenere un comparto che, anche a fronte di un costante abbattimento degli organici, offre sempre una tenuta non solo di grande efficienza, come ho detto, ma anche di emblematica dignità. Se la sicurezza costituisce una priorità nel programma di Governo, allora è necessaria un'azione di lungo respiro che, concertata e condivisa anche trasversalmente, possa effettivamente declinare serenità ed ottimismo degli addetti, da un lato, e credibilità politico-istituzionale dall'altro. Una strategia, onorevoli colleghi, che, abbandonando la pratica minimale della elargizione, della elargizione, peraltro insignificante, dell'*una tantum*, coltivi la cultura dell'azione sistemica, anche di medio e lungo periodo, contemplando interventi coerenti in termini non solo di riordino delle carriere e di benefici economici, ma anche di rivisitazione degli organici, di politica alloggiativa residenziale agevolata, di razionalizzazione delle competenze, delle strutture e del sistema tecnologico, che peraltro offre, nei tempi moderni che viviamo, grandi opportunità di coordinamento, seppure in un'ottica di riequilibrio della spesa. In definitiva, una strategia che, sconvolgendo la cultura tradizionalistica, consideri la sicurezza non più un costo, ma un vero e proprio investimento, nell'interesse della collettività tutta. Onorevoli colleghi, ho avuto il privilegio di operare in vari ruoli nel comparto Sicurezza per oltre quarant'anni, e quanto ho affermato promana proprio dal dato esperenziale di lunghissimo corso, ed auspico, da parte del Governo e dell'intero Parlamento, una migliore attenzione alla priorità sicurezza ed il più chiaro rispetto per gli uomini e le donne del comparto stesso. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'affrontare alcune delle ragioni a sostegno del provvedimento oggi all'esame, mi si consenta una breve ricostruzione della vicenda. Ebbene, con la conversione in legge del decreto-legge n. 78 del 2010, recante rigorose «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» Governo e maggioranza scelsero - con lungimiranza e una certa dose di innegabile coraggio - di legiferare sul contenimento della spesa connessa al pubblico impiego. Fu allora inevitabile chiedere un sacrificio a quel settore, che occupa circa un terzo dei dipendenti della pubblica amministrazione, ovvero i comparti Sicurezza e Difesa, e introdurre anche per chi vi opera il blocco per tre anni delle retribuzioni stipendiali ai valori del 2010. Un sacrificio al quale Forze di polizia, Forze armate e Vigili del fuoco non si sono sottratti, continuando a svolgere il proprio delicato lavoro con immutato senso di responsabilità e - mi si conceda - con immutato senso delle istituzioni. Ed allora, in occasione del prolungato passaggio parlamentare del disegno di legge governativo sul «collegato lavoro» (convertito con la legge 4 novembre 2010, n. 183) fu il Popolo della Libertà ad introdurre una fondamentale modifica al testo. Si volle infatti riconoscere la specificità la specificità del ruolo del comparto sicurezza per i «peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti», rimandando poi, in maniera esplicita, a «successivi provvedimenti legislativi» per lo stanziamento delle occorrenti risorse finanziarie. Stanziamenti che sarebbero dovuti transitare sul fondo, appositamente istituito all'articolo 8, comma 11-*bis*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, già destinato «al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco». e lo dico ai colleghi dell'opposizione - che in quell'occasione il PD si astenne dal voto sull'introduzione della connotazione di specificità, parlando di «norma manifesto», così come ricordo l'incredulità di alcune associazioni di categoria di fronte al plauso, pressoché generale, espresso dagli stessi addetti del comparto. Oggi - nei limiti dei ristretti margini di manovra concessi dalle misure di contenimento del *deficit* pubblico - il Governo intende compiere un primo passo per ripagare la fiducia accordatagli. E lo fa dando concretezza ai propositi espressi all'articolo 19 del «collegato lavoro» con lo stanziamento di 345 milioni di euro in tre anni, come si legge all'articolo 1 del decreto al nostro esame. Somma che, aggiungendosi ai 160 milioni di euro già disponibili sul predetto fondo, consentirà di erogare 195 milioni di euro per i primi due anni (2011 e 2012) e 115 milioni nel terzo anno. Una cifra che permette, soprattutto, di realizzare l'obiettivo di controbilanciare gli effetti del blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo e degli aumenti stipendiali nel periodo 2011-2013. va inoltre considerata positivamente la possibilità, configurata al comma 2 dell'articolo 1, di una successiva integrazione del fondo perequativo mediante la più snella procedura dell'atto amministrativo, in luogo della modifica per via legislativa, anche se il fatto che gli ulteriori stanziamenti a favore del fondo saranno conseguenti ad eventuali riduzioni della spesa per le missioni internazionali di pace pone obiettivamente la necessità di ricercare soluzioni di insieme che che esulino dal singolo conferimento di un contributo *una tantum*; ciò, anche perché la pratica di un incremento della dotazione del fondo perequativo, autorizzata dal comma 2 dell'articolo 1, apre inevitabilmente la strada al superamento stesso della logica dell'*una tantum*. Debbo infine sottolineare, come particolarmente degna di attenzione per i profili di interesse della Commissione difesa, alla quale appartengo, la composizione della copertura finanziaria, realizzata al comma 4 dell'articolo 1 con una riduzione degli stanziamenti previsti allo scopo del riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate e di polizia. È, questa, una disposizione che dovrà andare di pari passo con l'indicazione di un preciso indirizzo governativo, vista la rilevanza della materia per l'intero comparto Difesa e Sicurezza. Certo, a questo provvedimento non si può chiedere respiro progettuale, perché è soprattutto un intervento urgente che punta a sanare una condizione di sofferenza sociale, assegnando risorse, sia pur *una tantum*, ad un comparto che ha sempre dato prova di abnegazione e sacrificio. E a tal proposito, signor Presidente, mi consenta di ringraziare ancora una volta le Forze armate, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'opera che svolgono, quotidianamente, con ammirevole dedizione ed estrema professionalità, nell'intento di garantire la difesa del Paese e la sicurezza e dei cittadini. E lo dico senza retorica, perché così è veramente. Vorrei perciò concludere chiedendo al Governo, la cui sensibilità in materia è nota, un impegno per il futuro: al fine di rivedere - allo scadere del blocco del livello retributivo imposto alla pubblica amministrazione dalla vigente normativa - il concetto di elargizione *una tantum* là dove si legifera sulla condizione lavorativa

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,

dovrebbero essere destinate ad andare in economia ove non utilizzate, secondo un principio generale di contabilità pubblica. In relazione agli emendamenti esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.102 e 1.104, di semplice contrarietà sulla proposta 1.105 e di nulla osta sulle restanti proposte».

di venire in Aula, così come chiesto da tutti i Gruppi parlamentari di opposizione in più di una Conferenza dei Capigruppo, per aprire una discussione sui risultati e fare un bilancio di questi primi tre anni di politiche della sicurezza del Governo Berlusconi, con riferimento ad una serie di fatti specifici che hanno caratterizzato anche il ruolo internazionale del nostro Paese. Mi riferisco alla vicenda dei migranti dal Nordafrica e del del riconoscimento della protezione temporanea a 25.000 tunisini e alla bocciatura da parte della Corte di giustizia europea del reato di immigrazione clandestina; mi riferisco a più di una pronuncia della Corte costituzionale sulla illegittimità dei poteri sindacali in materia di sicurezza e quindi al fallimento delle cosiddette ronde; mi riferisco alla sentenza della Corte costituzionale, che ha dichiarato "esilarante dal punto di vista giuridico l'aggravante della clandestinità per quanto riguarda le condotte illecite. Mi riferisco tutte quelle bandierine ideologiche che il Governo e la maggioranza in questi tre anni hanno posto sui vari pacchetti sicurezza, senza ascoltare alcun consiglio dell'opposizione, e che sono state smontate dalla Corte costituzionale dalla Corte di giustizia europea e che comunque non hanno prodotto alcun effetto pratico, al punto che il Presidente del Consiglio è stato costretto a scrivere scrivere una lettera, insieme al presidente Sarkozy, nella quali i due *leader* si sono impegnati a rivedere l'Accordo di Schengen. accordo, così come previsto e attuato negli Stati membri dell'Unione europea, certamente con i limiti che l'Unione europea ha in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, determina sostanzialmente la circostanza che ciascun Paese deve farsi carico comunque del fenomeno migratorio. La lettera e l'iniziativa congiunta italo-francese è servita solo a dare una mano a Sarkozy nei confronti dell'Italia per la chiusura della frontiera con la Francia. Avremmo voluto cioè conoscere, anche di fronte a una serie di dichiarazioni improvvide del ministro Maroni e di altri autorevoli esponenti del Governo sulla Corte costituzionale, sulla Corte di giustizia europea e su tutto ciò che abbiamo letto sui giornali in queste settimane e in questi mesi, i risultati concreti conseguiti in i risultati concreti conseguiti in materia di sicurezza, di lotta alla clandestinità, all'immigrazione irregolare, e così via,

che credo sia esattamente la prova provata dell'oltraggio e della presa in giro nei confronti di poliziotti, carabinieri, rappresentanti della Guardia di finanza e di tutti coloro i quali si impegnano quotidianamente per garantire la sicurezza pubblica nazionale. I I nostri emendamenti, signor Presidente (di questo avremmo voluto discutere con il ministro Maroni ed il Governo), segnalano semplicemente la circostanza che nel provvedimento non vengono stanziate risorse aggiuntive per riconoscere la specificità del ruolo, della funzione e della professionalità delle Forze di polizia e del comparto sicurezza. Attraverso una sorta di partita di giro si rimpingua infatti un fondo sottraendo risorse al fondo previsto per il riallineamento delle posizioni di carriera del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e, per altro verso, al fondo fondo previsto già dal 2004 per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Si prelevano, cioè, risorse da questi fondi, che puntano a finanziare il riordino delle carriere del personale del comparto sicurezza, e si dà un un contributo *una tantum*, un obolo, una piccola elemosina di circa 24 euro mensili al personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, eccetera spacciando questo intervento per un provvedimento in favore del comparto e a presidio della sicurezza.

cosa sarebbe successo se questo Governo non avesse introdotto una sanatoria per 25.000 migranti provenienti dalla Tunisia! Avremmo avuto 25.000 processi in corso che avrebbero aggravato il già triste bilancio della giustizia italiana. Avremmo voluto parlare in tale circostanza, signor Presidente, anche dei provvedimenti, altrettanto demagogici, relativi alla immediata espellibilità degli extracomunitari reclusi condannati ad una pena superiore a due anni per capire, visto che per cento della popolazione carceraria è composta da extracomunitari e stranieri, se quei provvedimenti, tanto sbandierati nelle diverse campagne elettorali, fossero stati attuati, in che misura e che effetto deflattivo avessero avuto sulla situazione della popolazione carceraria italiana. Di tutto questo e di tutte le altre "bufale" che in questi tre anni ci avete rifilato avemmo voluto parlare con serenità nella sede propria, che è il Parlamento. Ci è stato risposto dal ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Vito, che il ministro Maroni ritiene di chiudere questa pratica che riguarda la sicurezza con l'ennesima routinaria, burocratica informativa al Comitato Schengen.

sull'immigrazione irregolare, sulle espulsioni effettuate realmente, su quelle con accompagnamento alla frontiera, su quante unità di personale vengono utilizzate nei centri e su quanti sono i centri di identificazione. che ci venisse a dire esattamente e con concretezza, e non a chiacchiere, cosa si è fatto e cosa si sta facendo, perché il silenzio conferma solo il fallimento, anche anche in questo settore, delle politiche del Governo Berlusconi. Per questo abbiamo presentato emendamenti che puntano, in questa fase, a trasformare un obolo *una tantum* in un

pensare di rimpinguare ulteriormente questo fondo diminuendo le risorse per le missioni internazionali (un altro modo indiretto di delegittimare i militari impegnati nelle missioni internazionali di pace all'estero), di tagliare drasticamente il finanziamento delle cosiddette auto blu limitandone l'uso solo ed esclusivamente alle esigenze di servizio di una cerchia ristretta e predeterminata esattamente

finestra"). È in tribuna una rappresentanza di studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Trapani. A loro va il saluto dell'Assemblea.

Presidente, colleghi, vorrei fosse chiaro a tutti che oggi siamo stati convocati per partecipare, in veste di comparse, ad uno *spot* elettorale, l'ennesimo, fortemente voluto dal Presidente del Consiglio che, come di consueto, nega la realtà e preferisce nascondere la polvere sotto il tappeto, anziché toglierla. Questo *spot* ritrae un Governo del fare, che si mostra estremamente sensibile alle istanze mosse dalle Forze armate e dalle Forze di polizia e di sicurezza e che decide di dare loro un premio per l'encomiabile e fondamentale lavoro svolto, attraverso il riconoscimento di un compenso economico. una favola a lieto fine in cui il personale del comparto viene premiato dal buon amministratore. La realtà è ben diversa. Quanti hanno fino ad oggi operato per garantire la sicurezza al Paese diventano, per l'ennesima volta, vittime di un raggiro. Entrando nel merito del provvedimento, a determinare l'urgenza del decreto-legge n. 27 del 2011 è stato innanzitutto un fattore: si è ravvisata la necessità di porre rimedio

Con tale atto normativo, nello specifico con l'articolo 9, commi 1 e 21, il Governo aveva deciso di far fronte alla crisi economica, che il Presidente del Consiglio ha sempre negato, attraverso l'introduzione del blocco degli effetti economici delle promozioni. In breve, si è deciso di non incidere sulle strutture gerarchiche che caratterizzano le Forze armate e di polizia, di non bloccare le promozioni e gli avanzamenti di grado, ma semplicemente di non riconoscere i trattamenti economici fino al 2010 previsti per tali avanzamenti. di metafore - «la botte piena e la moglie ubriaca». Il personale del comparto ha comunque accettato questa decisione e ha continuato a svolgere egregiamente il proprio dovere. I tenenti promossi hanno assunto la responsabilità dei capitani e hanno iniziato a svolgere le nuove funzioni senza però aver ottenuto un incremento nel trattamento economico. Lo hanno fatto sicuramente perché hanno un fortissimo senso del dovere, di cui siamo tutti grati. Ma fino a che punto questo Governo intende fare leva su tale sentimento? Quante altre prove di pazienza saranno costrette a sostenere le Forze di polizia e quelle dell'ordine? Questo decreto-legge rappresenta sicuramente l'ennesima prova cui viene sottoposta la pazienza del comparto Difesa. Come possono le Forze addette a garantire la sicurezza del Paese sentirsi appagate dal riconoscimento di un assegno *una tantum*, di valore sicuramente molto esiguo? Ma il problema, colleghi, non proviene solo dai criteri adottati per gestire tali risorse; a preoccuparci è soprattutto la copertura che il Governo ha deciso di dare a tale decreto-legge, a tale grandissima, incisiva e soprattutto lungimirante manovra politica, comprese le conseguenze che ne derivano. Gli assegni *una tantum* che verranno corrisposti al personale delle Forze armate e di polizia ai vigili del fuoco saranno versati attingendo completamente dal capitolo «riordino delle carriere e riallineamento dei ruoli». La promessa fatta dal Governo ad inizio legislatura di riordinare le carriere e di dare maggiore dignità alle forze di sicurezza, anche attraverso un trattamento economico più favorevole, viene, quindi, attraverso questo decreto-legge, completamente spazzata via. Il Governo, da oggi, non avrà più i fondi per affrontare questi due importantissimi aspetti della questione. Possiamo chiudere definitivamente nel cassetto il sogno di riordinare le carriere e i ruoli del personale dei comparti sicurezza e difesa. Sempre in tema di copertura, il Governo ha deciso di assicurare un eventuale ulteriore finanziamento del fondo di cui al comma 1 attingendo anche dal fondo delle missioni internazionali. Il Governo, infatti, prevede inspiegabilmente di destinare minori risorse in campo internazionale rispetto agli anni precedenti. Questa previsione di spesa risulta, però, ingiustificata, soprattutto alla luce dei nuovi drammatici sviluppi in Medio Oriente e nel Nord Africa a partire dalla missione in Libia, e della costante esiguità delle risorse storicamente destinate Inoltre, gli stanziamenti previsti, secondo il Governo, potrebbero anche essere incrementati utilizzando i fondi derivanti dai risparmi delle altre amministrazioni dello Stato! Vorrei complimentarmi, dunque, con le altre Amministrazioni dello Stato. I miei complimenti vanno al Ministero dei beni e delle attività culturali che, nonostante la drammatica situazione in cui versano le opere d'arte, riuscirà a risparmiare. Vorrei inoltre elogiare il Ministero dell'istruzione che, nonostante i problemi di organico e le emergenze strutturali degli edifici scolastici, riuscirà anch'esso a risparmiare. Vorrei infine complimentarmi con il Ministro della salute che nonostante l'elevatissimo numero di ricoveri ospedalieri e la carenza strutturale e organica, dovuti alla politica del taglio indiscriminato adottata da questo Governo, riuscirà, risparmiando, a finanziare il fondo e a garantire che le forze dell'ordine percepiscano una irrisoria somma *una tantum*. Occorre inoltre dire che tali eventuali incrementi del fondo verranno disposti con decreto ministeriale, bypassando le consuete procedure di verifica parlamentare sugli aspetti finanziari. In pratica, quindi, si permette al Ministro dell'economia e delle finanze di diventare l'esclusivo gestore delle risorse nazionali, eludendo qualsiasi possibile interferenza da parte del potere legislativo, costituzionalmente atto atto a svolgere una funzione di vigilanza. Concludo, colleghi, annunciando il voto di astensione del mio Gruppo. Abbiamo deciso di non opporci, esclusivamente perché sarebbe un'ulteriore ingiustizia nei confronti di quanti lavorano nei comparti Difesa e Sicurezza, negare persino questo piccolissimo atto di elemosina che il Governo ha inteso compiere. Sicuramente, se fossimo stati noi al governo, non saremmo stati costretti ad adottare tali vergognose misure riparatrici, ma avremmo messo in atto una politica di lungimiranza e di efficienza, che è ben lontana dalla realtà che ormai tristemente contraddistingue l'agire di questo Esecutivo.

tuttavia, ci troviamo di fronte ad un primo importantissimo gesto concreto in favore dei nostri uomini che difendono la legalità e la democrazia in Italia come all'estero. Il comparto Sicurezza e Difesa è il primo - e ad oggi l'unico - di tutto il pubblico impiego a ricevere e ad incassare un concreto provvedimento legislativo di natura economica: certo, solo sulla base stipendiale (che ha subito un blocco) di questi uomini, non sulle parti accessorie e sugli straordinari, però incontrovertibilmente stiamo parlando di una nuova disponibilità finanziaria per il comparto stesso, peraltro come prima e unica eccezione al decreto-legge n. 78 dell'anno scorso, più volte citato durante la discussione generale, con riferimento alla specificità di questo settore, che viene ampiamente riconosciuta dal Governo. Alle nostre Forze armate e di polizia e ai Vigili del fuoco destiniamo un aumento quando altri Paesi europei si sono trovati costretti addirittura a licenziare decine di migliaia di appartenenti per far quadrare i bilanci, come in Gran Bretagna, dove circa 30.000 poliziotti sono stati licenziati. Purtroppo, la congiuntura economica ci permette per ora di aggiustare il tiro e far fronte solo in parte agli eccessi dei tagli lineari che questo comparto aveva subito, come tutti gli altri settori pubblici,

che prevede come prima destinazione proprio il supporto economico alle forze di sicurezza, anche tramite l'assegnazione di somme *una tantum*, come stabilito dalla finanziaria del 2010. Appare pertanto strumentale anche solo affermare che il Governo «aumenta di 25 euro al mese lo stipendio ai poliziotti», perché le assegnazioni non saranno a pioggia, ma saranno elargite a chi ha subito effettivi tagli o blocchi sull'avanzamento del compenso, con particolare riferimento all'anzianità di servizio, partendo infatti da chi ha almeno 17 anni di servizio. Va poi specificato che il testo del decreto-legge deliberato dal Consiglio dei ministri prevedeva due diverse forme dell'eventuale integrazione del Fondo, una per il personale del comparto difesa e una per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Più precisamente, il testo del Governo prevedeva che potesse essere destinata solo al personale delle Forze armate una parte dei risparmi corrispondenti alle eventuali minori spese effettuate rispetto al precedente anno per missioni internazionali di pace, mentre al personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco potessero essere destinate risorse eventualmente disponibili nel Fondo unico per la giustizia. Le modifiche apportate alla Camera, con la disponibilità anche in questo caso del Governo, hanno voluto, da una parte, eliminare tale rigidità nella destinazione delle risorse disponibili sui due predetti Fondi, quello per le missioni internazionali di pace e quello del Fondo unico, e, dall'altra, prevedere un ulteriore canale di finanziamento eventuale delle misure in favore del personale dei comparti Difesa, Sicurezza e Protezione civile, prevedendo la possibilità di utilizzare

dei tre comparti non impegnate nell'esercizio di competenza possano essere utilizzate per i medesimi scopi nell'anno successivo, anche aggiungendosi alla dotazione prevista per il nuovo anno. anno. Il comma 3 è stato poi modificato al fine di specificare che gli assegni al personale sono assegni perequativi individuali, aventi la stessa natura giuridica dell'emolumento corrispondente, e non soltanto assegni *una tantum*, come prevede il testo base del Governo. Ci sembra che tali modifiche siano state quanto mai opportune per dare più equilibrio ed equità ai vari corpi del comparto. Ovviamente, è necessario che il Governo si impegni, come ha fatto in Commissione accettando l'ordine del giorno firmato anche dal mio Gruppo e a prima firma del collega Saltamartini, che ringraziamo,

propositivo al disegno di legge in esame, ma con la volontà di verificare gli altri impegni del Governo per questo comparto. Presidente, rileggendo i provvedimenti sottoposti al Parlamento dal Governo negli ultimi mesi - penso al processo breve, a quello definito lungo, ai vari impedimenti, legittimi o meno veniva da credere che difficilmente se ne sarebbero potuti registrare di peggiori. Ma poi è arrivato questo decreto-legge, che assegna un obolo alle Forze armate, alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco. Si affronta cioè la drammatica situazione del settore: mettendo in campo una misura *una tantum*. È questa la dimostrazione di quanto il Governo, al di là della propaganda quotidiana, tenga effettivamente alla sicurezza, di quanto tenga alle Forze armate, oltre che chiamare quotidianamente chi vi opera «i nostri ragazzi», o alle Forze di polizia, salvo poi vantarsi di arresti e sequestri in campo mafioso. Desidero sottolineare una volta per tutte, dato atto al ministro dell'interno Maroni, al quale va la mia incondizionata stima, di aver proposto una legge sacrosanta, peraltro sostenuta ed approvata da tutti,

Potrei stilare un elenco infinito, a cominciare da Riina, Provenzano, Madonia, Schiavone, Vernengo, Santapaola, e così via. Ognuno di questi è il risultato dell'attività ininterrotta, oltre che della magistratura, oggi tanto vituperata, soprattutto delle Forze dell'ordine, alle quali va il riconoscimento del Governo che le premia - udite udite - con un obolo. Eppure, l'Esecutivo sa bene che non si tratta di questioni meramente economiche, ma di argomenti che investono la specificità del lavoro, i contratti, il blocco degli stipendi, la previdenza, il riordino. Il Governo è stato solo abile. Ma dove vive? In quale realtà vive? Non si rende conto che è riuscito a coagulare tutti i sindacati, tutte le organizzazioni sindacali, vicino al pensiero di destra, vicino al pensiero di sinistra tutte - nella contestazione per riaffermare i propri diritti. E quando gli agenti hanno raggiunto la residenza di Arcore del Presidente del Consiglio, lo stesso Presidente è sceso tra i manifestanti garantendo il suo personale intervento e lo stanziamento al successivo Consiglio dei ministri

si tratta di 340 milioni di euro in tre anni. aa parte che l'ultimo anno è tutto da discutere, egli probabilmente non si è reso conto

considerati gli spaventosi tagli degli ultimi tempi. Inutile è stato allora il tentativo di tradurre il trattamento compensativo *una tantum* con un altro fisso, continuativo, valido ai fini pensionistici. Eppure, il consenso intorno a questa soluzione era stato raggiunto in Commissione alla Camera dei deputati fino al consueto passo indietro dell'Assemblea, prona ad ogni espressione di volontà del Governo. Mi chiedo allora fino a che punto si abuserà della pazienza degli uomini e delle donne che rischiano quotidianamente - quelli sì - la vita per salvare la collettività e con il loro lavoro consentono ad esponenti dell'Esecutivo di affacciarsi costantemente in televisione per proclamare arresti e sequestri. Fino a quando i nostri militari impegnati in missioni di pace affronteranno gli attacchi proditori di chi quella pace non la vuole, sentendosi inoltre penalizzati e offesi da un provvedimento simile? Quando si parla di Forze armate, di Forze dell'ordine e di Vigili del fuoco - di questi ultimi, colpevolmente, troppo poco ci si occupa - lo facciamo con orgoglio. Siamo consapevoli del loro ruolo fondamentale e siamo coscienti che certe razionalizzazioni si devono compiere riducendo sprechi, duplicazioni di funzioni e di ruoli, ma siamo altrettanto consapevoli che è indispensabile garantire le risorse per mettere la Difesa e la Sicurezza al riparo dalle congiunture economiche. Non c'è, in definitiva, soltanto un problema di rivendicazione salariale. La questione dell'*una tantum* finisce per mortificare l'intero settore, come mortificante è il fatto che le risorse debbano essere raccattate qua e là, come se si trattasse di una elargizione, probabilmente solo in risposta alle manifestazioni di protesta degli agenti. Disporre un obolo significa non voler affrontare e risolvere i problemi che meritano una impostazione di carattere generale, soprattutto per quanto attiene agli avanzamenti, alle carriere e alla previdenza. L'Esecutivo non ha capito, o non vuole capire, che, oltre l'esigenza di una soddisfazione materiale, una grande frustrazione da parte di quegli uomini delle Forze dell'ordine, costretti a lavorare in zone notoriamente a rischio e non supportati dagli strumenti più elementari.

può vedersi anche attribuita un'elemosina di 23 euro; ma costui vorrebbe poter svolgere il proprio lavoro con serietà, professionalità e dedizione e vorrebbe essere messo in condizioni di contare su uomini e mezzi. Mi chiedo: il Governo pensa veramente di chiudere la partita con questa donazione? Se l'Esecutivo è convinto di questo, ne resto sconvolto, ma prenderò atto che il tema del comparto Sicurezza viene affrontato solo per motivi elettorali e - quindi - di consenso. Per questa ragione, dichiaro che il mio Gruppo si asterrà. È un'astensione che suona come una presa di distanza dalla politica di questo Governo che, in una visione miope e marginale delle reali difficoltà, vorrebbe risolvere il problema in un modo a dir poco umiliante. Con il nostro voto di astensione vogliamo difendere i principi e i valori di cui sono portatori i destinatari del provvedimento e non dare la nostra adesione alla politica della sicurezza dell'Esecutivo. *(Applausi

e onesti: dobbiamo assolutamente dire che il voto di astensione in Senato non è tale, ma è un voto contrario, per cui ci si sta mascherando dietro una cosa che non è vera.

le forze di polizia ci consentano di andare in televisione a fare degli *spot* elettorali, perché il ministro Maroni e tutti gli uomini cercano di dare il massimo per assicurare alle

con il voto finale in Aula al Senato è emblematica, colleghi della maggioranza, della vostra assoluta incapacità di governare in modo serio e credibile questo nostro Paese.

a piazza del Popolo, in occasione del 150º anniversario dalla fondazione del Corpo della Polizia di Stato, annunciò con grande coraggio e anche con assoluta buona fede, ne sono convinto, che si sarebbe avviata immediatamente la riforma dell'ordinamento della pubblica sicurezza in Italia.

aveva non solo dichiarato la propria disponibilità, ma addirittura sollecitato un intervento di riforma organica del settore, tanto che la Commissione affari costituzionali - il collega Vizzini lo ricorderà certamente

Lo stesso identico approccio, colleghi della maggioranza, lo avete avuto per quanto riguarda la questione della polizia locale. La Commissione affari costituzionali ha varato, tra l'altro in modo condiviso, un testo di riforma che riguarda un settore delicato quale quello della polizia locale. Questo provvedimento, praticamente pronto, e che ha due relatori, uno nominato tra le forze di maggioranza e uno tra le forze di opposizione, è fermo perché il Governo non dà via libera dal punto di vista della copertura finanziaria, peraltro estremamente ridotta. Insomma, io credo Insomma, io credo che voi affrontiate una questione delicata ed importante in un modo assolutamente inadeguato. Vi è sofferenza, colleghi, tra le Forze di polizia e Forze armate.

La politica complessiva del Governo in questa materia naturalmente non ci può soddisfare. Ci sono certamente sprechi in un settore delicato, ma non ci sono risorse adeguate per quegli uomini e donne delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle Forze armate che fanno il loro dovere in modo così appropriato e che soffrono di una condizione difficile, nelle frontiere sia militari sia di sicurezza in cui sono quotidianamente impegnati. Ed è a loro che noi affidiamo sistematicamente la difesa del nostro Paese in in situazioni molto delicate, e li ripaghiamo con un obolo, colleghi. Ha ragione il collega Serra: si tratta di un obolo vergognoso, di una cifra incredibile, di 23 euro lordi, e per di più - lo voglio dire al collega Torri che si lamenta perché le forze dell'opposizione hanno deciso di astenersi astenersi - avendo rigettato qualche attimo fa gli emendamenti che almeno trasformavano un obolo in un assegno permanente e non *una tantum*.

vi riempite la bocca dei successi delle Forze di polizia o della qualità dei nostri uomini delle Forze armate e poi, al momento giusto, dimenticate di premiare la loro professionalità e di lavorare in questa direzione. Ecco la ragione per la quale non possiamo in questa condizione che dissociare la nostra responsabilità dalla vostra. Naturalmente noi non voteremo contro, proprio per rispetto delle Forze di polizia e perché la loro condizione di malessere è tale che anche una goccia va difesa. Ma ci impegneremo con tutte le nostre forze, a partire dalla ripresa dell'attività parlamentare, per una vera riforma dell'ordinamento della pubblica sicurezza e perché sia pagata in modo adeguato la professionalità che noi richiediamo a questi uomini. Per questa ragione i senatori del Partito democratico non voteranno per questo provvedimento e si asterranno, come gesto di attenzione e di rispetto nei confronti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, negli ultimi 15 anni il nostro Paese è stato governato per otto anni dal centrodestra e per sette anni dal centrosinistra. Nel quinquennio 2001-2006 il Governo Berlusconi finanziava la legge sui parametri con 530 milioni di euro e la contrattazione collettiva e la specificità con 1 miliardo e 690 milioni di euro. Nel successivo biennio il Governo di centrosinistra, guidata dal presidente Prodi, incrementava la tassazione del personale dipendente pubblico, portando l'aliquota dal 23 per cento al 27 per cento. Con la crisi finanziaria internazionale che voi conoscete, affrontata con il decreto-legge n. 78 del 2010, nel pubblico impiego si sottoponevano ad una sterilizzazione tutti i trattamenti contrattuali del personale del pubblico impiego. E tuttavia, dopo una lunga rivendicazione di questo personale, che sottolineava come il proprio ordinamento, lo stato giuridico, e conseguentemente il trattamento che ad esso doveva essere riservato in base all'articolo 36 della Costituzione dovesse essere

ad approvare la legge sulla specificità, con l'articolo 19 del collegato al lavoro entrato in vigore nell'ottobre dello scorso anno. La legge sulla specificità non è affatto quanto è stato sostenuto in quest'Aula. C'è un principio che voi, colleghi della sinistra, probabilmente potete sostenere: il principio di uguaglianza dei trattamenti dei dipendenti pubblici. Impossibile immaginare che si possano riconoscere trattamenti privilegiati. Ebbene, con le norme sulla specificità sosteniamo la tesi che questo personale, che non esercita i diritti di rappresentanza come tutti gli altri lavoratori, che non ha i diritti politici come tutti gli altri cittadini, deve ottenere uno *status* che ne riconosca le peculiarità le peculiarità attraverso riconoscimenti normativi specifici. Se mi è consentito, dopo trent'anni che tale rivendicazione andava avanti, questo è il primo provvedimento in cui si riconosce a detto personale che le sue prestazioni non sono esattamente uguali a quelle degli altri pubblici dipendenti. Per essere concreti, sottolineo che chi ha letto questo provvedimento non ve lo ha spiegato bene. Non è vero che gli aumenti sono pari a 23 euro lordi a testa: gli incrementi retributivi sono parametrati sui trattamenti specifici e riguardano l'assegno di funzione, la parametrazione, le promozioni, le classi e gli scatti dei dirigenti PdL),* gli aumenti ISTAT dei dirigenti. E per dare dei numeri (non i numeri al lotto), per il personale con 17 anni di servizio appartenente al ruolo degli agenti, sovrintendenti e ispettori

per il personale con 27 anni di servizio il provvedimento riconosce 1501 euro lordi l'anno; per il personale con 32 anni di servizio riconosce 343 euro lordi l'anno a solo titolo di assegni funzionali. Quindi, cari colleghi presenti, non credo che questo personale possa essere strumentalizzato da una parte o dall'altra attraverso la demagogia. Quando siete stati Quando siete stati al Governo non avete riconosciuto i benefici che oggi sostenete; mi auguro che quando andrete al Governo possiate farlo, ma finora non l'avete fatto. Veniamo ora alla questione del trattamento e del riordino delle carriere.

Ricordo in quest'Aula che, nel 2006, un progetto di legge di riordino delle carriere, che avevo contribuito a redigere, fu approvato fu approvato dalla Camera dei deputati e poi, per una serie di problemi, non fu approvato dal Senato della Repubblica. Mi auguro che in questa legislatura potremo

queste misure sono dovute agli uomini che garantiscono l'ordine pubblico internazionale all'estero e nel nostro Paese. Questi trattamenti sono dovuti a chi garantisce la lotta alla mafia e alla criminalità organizzata e i servizi di ordine pubblico.

quindi orgoglioso di dichiarare oggi (domani è la Festa della Polizia) che il Governo Berlusconi, nonostante la crisi internazionale e il blocco delle retribuzioni, riconosce a tutti gli appartenenti al personale delle Forze armate e delle Forze di polizia il ruolo e lo *status* che a loro spetta, in funzione della loro attività loro attività e del rischio della vita, che molto spesso corrono nello svolgimento dell'attività istituzionale. Questi sono fatti. La demagogia spero sia abbandonata alla campagna elettorale, che spero possa terminare domenica prossima. *(Applausi

alla votazione finale di questo provvedimento perché sono state formulate in questa Aula delle affermazioni gravissime nei confronti dei confronti dei senatori del Partito Democratico. Cominciamo dalla specificità: invito il senatore Saltamartini ad andare a ricercare il disegno di legge del 18 settembre 2008

Forze armate e che era sottoscritto da tutti i parlamentari del Partito Democratico: esso prevedeva il riconoscimento della specificità per le Forze dell'ordine, le Forze di Polizia e le Forze armate. Sono state poi fatte altre affermazioni errate. Naturalmente nell'ambito del Partito Democratico operano personale e senatori che conoscono perfettamente quali sono le motivazioni e l'impegno dei nostri uomini e delle nostre donne delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco. Quindi, credo che quelle affermazioni che sono state formulate in quella circostanza siano state assolutamente fuori luogo ed errate. Per questo non parteciperò alla votazione*.

con ricorso depositato il 14 dicembre 2010, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in relazione alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 21 aprile 2010, ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadevano, pertanto, nell'ipotesi di immunità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. (*Doc*-*IV*-*ter*, n. 14). Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 6 aprile 2011, n. 142, depositata in cancelleria il successivo 15 aprile e notificata al Senato il 6 maggio 2011. Nella seduta del 17 maggio 2011 la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

colleghi, sull'atto principale che dobbiamo ricordare in questa seduta, e cioè se l'attività giornalistica dell'ex senatore Iannuzzi fosse un'attività parlamentare o se fosse la sua attività professionale, il Gruppo del Partito Democratico, molto liberamente ma molto unitariamente, ha ripetuto credo almeno una quindicina di volte in questa legislatura che di attività giornalistica si trattava e non di attività parlamentare. Oggi ce lo ricorda anche il tribunale di Milano, che sottopone al giudizio della Corte costituzionale il fatto che il Senato, come tante altre volte su casi come questo, sbaglia nell'applicare le disposizioni costituzionali. siccome non siamo malati di coazione a ripetere e a ripetere le brutte figure del Senato davanti alla Corte costituzionale, per semplice salvezza - diciamo così

costituiamoci nelle forme previste dagli articoli 20 e 37 della legge di procedura della Corte costituzionale (la legge n. 87 dell'11 marzo 1953) che prevedono l'intervento diretto, il privilegio dell'intervento diretto, e la comparsa personale degli organi dello Stato senza dare incarichi a professionisti del libero foro. Se questa clausola non fosse contenuta nella deliberazione del Senato, per evitare la brutta figura riteniamo che il Senato non si debba costituire in giudizio davanti alla Corte costituzionale nel conflitto di attribuzioni sollevato dal tribunale di Milano, un ricorso che perderemo senz'altro. LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo reiterando un rito. Dal 1992 siamo riusciti a perdere innanzi alla Corte costituzionale oltre il 95 per cento delle cause. Cioè, perdiamo sempre: ci danno sempre torto. Ci sarà un motivo per cui si perde sempre? Su 1.200 processi innanzi alla Corte costituzionale abbiamo perso circa 1.100 volte. Ma quanto ci è costato questo *record*? E visto che non possiamo arrivare matematicamente al cento perché non rinunziamo ad inseguire un *record* impossibile, considerando che ogni volta che partecipiamo a questa gara paghiamo

così granitica nella difesa delle cause perse, ritrovi allora un po' di ragione. non votiamo a favore di questo provvedimento perché ci sembra di aver superato la soglia del ridicolo.

pertanto autorizzata a conferire mandato per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato ad uno o più avvocati del libero Foro.